L’elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. decreti-legge». In data 29 gennaio 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro per le politi- che giovanili e lo sport: «Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)» (2077). In data 30 gennaio 2021 è stato presentato il seguente disegno di legge: dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro della giustizia: Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7, recante proroga di termini in materia di accertamento, riscossione, adempimenti e versamenti tributari,

«Sto pensando ai tanti invisibili della neve e, con umiltà, condivido il mio pensiero. In un mare di notizie, numeri, decreti e tanta incertezza, la montagna, dignitosa e silenziosa, sta passando un tragico invisibile inverno. Come una dama di infinita bellezza, vestita del suo abito bianco migliore, splendente e pronta come una sposa, non può donarsi ai tanti occhi e sorrisi che la vorrebbero ammirare ancora una volta. Tutto è immobile e tutto attende mentre un intero sistema economico, familiare, di equilibrio psicofisico ed emotivo sta scricchiolando e rischia di inabissarsi silenziosamente sotto il bianco della neve. La gente di montagna conosce il silenzio, non solo lo vive ma ne è parte integrante e ha un pudore innato. La gente di montagna convive con il freddo, le distanze e le grandi difficoltà per amore di un ambiente naturale che è ricevuto in dono e viene protetto e condiviso con coloro che sono da sempre graditi ospiti di questo territorio. La chiusura degli impianti sciistici, la chiusura degli alberghi, il mancato lavoro di maestri di sci, addetti stagionali degli impianti sciistici, di negozi, ristoranti, bar, cuochi, camerieri, addetti alle pulizie, tassisti, animatori, gruppi musicali, associazioni sportive e ogni altra attività connessa alle predette - ossia praticamente tutte - è uno scenario drammatico e toccante. Se infatti da un lato tutti comprendono e in gran parte accettano questo sacrificio per rispetto della situazione emergenziale del Servizio sanitario pubblico, il sentimento di sconcerto e in molti casi di disperazione sta prendendo il sopravvento per la pressoché totale mancanza, ad oggi, di un supporto economico concreto e consistente da parte dello Stato.

Signor Presidente, alcuni deputati in forza alla Lega hanno scritto un emendamento al decreto milleproroghe che così recita: «fino alla data del 31 dicembre 2025 la verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, 18 aprile 2016, n. 50, è necessaria solo per le aree soggette a specifica tutela negli interventi urbanistici. Per i casi non ricompresi nel precedente periodo è sufficiente l’autocertificazione di un progettista abilitato». Poiché lo strumento della verifica preventiva dell’interesse archeologico è riservato, nella normativa vigente, proprio alle aree non tutelate, si capisce bene chi siano i nemici giurati dell’archeologia preventiva. Del resto, la prossimità dei firmatari dell’emendamento a certi signori dell’eolico è notoria. Questo emendamento, che peraltro è in palese contraddizione sia con l’articolo 28 del codice dei beni culturali, sia con la Convenzione europea de La Valletta, ratificata anche dall’Italia, viene proposto in nome di un malinteso snellimento degli iter progettuali. In realtà, non solo indebolirebbe gravemente l’azione di tutela svolta dalle soprintendenze sul patrimonio archeologico, con conseguenze distruttive per tale patrimonio, ma rischierebbe persino di allungare i tempi e far lievitare i costi dei cantieri a danno esclusivo dei finanziamenti pubblici. La stessa direzione generale ABAP del Ministero, dopo la presa di posizione di tutti gli interessati, l’ha criticato pubblicamente. Presidente, detestare aggettivi come “amovibile” o “resiliente”, sostantivi come “valorizzazione” o “semplificazione” non per i concetti che esprimono naturalmente, ma per l’uso distorto e malsano che se ne fa, non basta più. Bisognerebbe bandirli dal linguaggio delle amministrazioni e del dibattito pubblico. È una provocazione la mia, naturalmente, ma non scherzo affatto quando dico che emendamenti come quello della Lega sono incostituzionali, se ancora vige l’articolo 9 della Costituzione, che recita: «La Repubblica (…) Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». O forse la parola «tutela» è stata bandita dal Paese